Nella maniera in cui è stato scritto a me sembra francamente forse pletorico, forse retorico, senz'altro esorbitante. Dice il comma 2 dell'articolo 2: «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta

Ha semplicemente una funzione stabilita dalla legge di tutelare il cittadino nella giurisdizione. Entrambi gli emendamenti, il primo in maniera più radicale,

L'emendamento 2.216 sarà valutato dal relatore e dal Governo. Asciuga il testo, ma in fin dei conti è quasi del tutto privo di portata normativa. Per questa ragione, me lo dico da solo, è al limite dell'inammissibilità. Invece, Invece, l'emendamento 2.217, senza modificare l'impianto stabilito dalla proposta che perviene dalla Commissione, propone di riordinare il testo, collocando nell'articolo 65, destinato ad essere articolo contenitore di tutte le norme transitorie, quel che succede con riferimento agli avvocati che si iscrivono agli albi dopo che sarà entrata in vigore questa legge e agli avvocati che già sono iscritti. Tuttavia, contiene una una prescrizione che a me sembra opportuna, che si legge nel secondo periodo della proposta. Mi riferisco a quella in cui si dice che per un periodo di tre anni gli avvocati già iscritti all'albo possono continuare la loro attività, così come finora l'hanno svolta, ma che dopo i tre anni dovranno rimuovere le eventuali incompatibilità, comprese quelle previste da questa nuova legge di riforma. L'emendamento 2.222 svolge una doppia operazione.

Non trovo assolutamente opportuna la parafrasi che il testo svolge rispetto alla norma costituzionale che riguarda i magistrati. Pur tuttavia, se la stessa si vuole mantenere, credo si debba farlo con il doppio intervento dall'emendamento: all'articolo 2, quando si parla dell'attività dell'avvocato; all'articolo 23, comma 3, quando si parla delle funzioni del Consiglio dell'ordine. L'emendamento 2.229 apre un tema assai complicato, su cui credo che il relatore e il Governo debbano soffermarsi anche per controllare l'armonicità dell'eventuale testo risultante con altre disposizioni di legge. L'emendamento propone di aggiungere i procedimenti di mediazione e di conciliazione alle attività esclusive dell'avvocato. Credo fermamente che il futuro dei 230.000 avvocati che oggi praticano la professione nel nostro Paese implichi per le future generazioni che l'avvocatura nella sua prospettiva sia articolata su un modello diverso dall'attuale, sotto pena di veder sempre più crescere il contenzioso civile e penale, senza vedere una fine a quella che è ritenuta, e giustamente è detta, la crisi della giustizia nel nostro Paese. Uno dei modelli possibili, il cosiddetto modello francese, vede un numero ristretto di avvocati patrocinatori davanti alle corti e un numero assai più ampio di quelli che i francesi chiamano i consulenti giuridici, cioè tutti coloro che assistono i cittadini dando le loro dando le loro prestazioni sia nella materia stragiudiziale sia nella sede della conciliazione e della mediazione che, come sappiamo, sono istituti da tempo conosciuti negli altri ordinamenti. Pur tuttavia, non è possibile introdurre un diverso modello di questo tipo, almeno a mio modo di vedere, senza misure di accompagnamento. Pertanto questa proposta, nella problematicità

del disegno di legge anche l'avvocato stabilito. Una volta che lo stesso esiste, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, deve essere ricompreso nelle specificazioni previste da questa norma.

Il testo presentato all'Assemblea è già un testo su cui la Commissione aveva accolto l'emendamento da me proposto durante l'esame in quella sede. 2.251 è una proposta di perfezionamento che vuole estendere al giurista d'impresa che lavora per un gruppo collegato di imprese la possibilità di svolgere il lavoro di consulenza per il proprio datore di lavoro o, meglio, per tutte quelle società raccolte raccolte nell'unico contenitore del suo sostanziale datore di lavoro. Quindi, è un ampliamento di possibilità.

che, ancorché abbiano origine da un avvocato, siano poi in concreto distribuiti da un soggetto diverso dall'avvocato e che non possa dunque esservi aggiramento della norma che impedisce

finestra"). Colleghi, è presente nelle tribune una delegazione dei componenti della Commissione agricoltura del Parlamento romeno, alla quale va il saluto dell'Aula.

intelligente e cortese, com'è nel suo stile, della collega Poretti che questa mattina, notando la mia assenza - della quale mi dolgo, anche se dovuta ad impegni politici esterni - si rammaricava per il mancato sostegno a tante iniziative comuni, come attestato dagli emendamenti

Federazione italiana giovani avvocati e dall'*Antitrust*, che abbiamo raccolto, sempre attraverso Internet, e che abbiamo ritenuto di condividere. Ho letto bene sul sito che l'ADUC aveva individuato in lei, nel senatore Ichino, nel collega Perduca e nella presidente Bonino gli interlocutori privilegiati di questa attività; ma il fatto che queste istanze fossero così ben rappresentate, non impedisce che altri, pieni di buona volontà ed intenzionati a far bene questo lavoro,

se c'è una filosofia che io contesto nel provvedimento del Governo, che ha sancito un patto evidente con la "corporazione" rispettabilissima e nobilissima dell'avvocatura italiana, è che, sul presupposto di una formazione inadeguata e di un accesso indiscriminato che determina la moltiplicazione del numero degli avvocati, si abbia un abbassamento della tecnica del diritto nel nostro Paese, con una scarsa qualità della professione. L'obiettivo però è molto diverso ed emerge da tutto il contesto del disegno di legge: si tratta di ridurre, in modo drastico il numero degli avvocati e garantire ai sopravvissuti, perlopiù anziani, di grande forza anche contrattuale nel rapporto con le giovani generazioni, introiti sempre più cospicui, che rafforzino la condizione di privilegio dei vertici professionali. Noi riteniamo invece che, in sintonia con le prescrizioni dell'Unione europea

debba essere stralciata la riforma della professione forense dal tema più ampio della riforma degli ordini professionali, considerato che, mentre in quel contesto si fa la scelta di una vasta liberalità e di una grande apertura, in questo caso invece, forse per la forza della "corporazione", che è un'antica tradizione italica che non viene mai meno, si impone al Parlamento di legiferare solo su questa materia per garantire il privilegio della «casta sacerdotale» degli avvocati.

in virtù delle capacità di convinzione che il senatore Pistorio ha manifestato nell'esprimere il motivo della sua adesione a determinati tipi di suggerimenti.

sapendo che chi farà proprio un emendamento, riuscirà, anche in virtù della qualità del lavoro svolto, a motivarlo. L'assenza era stata notata per la mancanza di sostegno a questo processo emendativo. L'articolo 2, in aggiunta alle attività già riservate, prevede di estendere l'esclusività della professione alle seguenti attività: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di conciliazione e mediazione (in particolare al comma 5 l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (in particolare al comma 6 dell'articolo l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati nel comma 7. I nostri emendamenti vogliono inserirsi in tutte queste specifiche competenze esclusive, cercando di riaprire, anche ad altri soggetti, la possibilità di prenderne parte. L'attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave, secondo noi, della concorrenza (più volte stigmatizzata dall'*Antitrust*), in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L'esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge. La restrizione, da un lato, comporta l'attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte e, dall'altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al potere economico della categoria titolare della riserva. L'ordinamento comunitario, però, pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l'osservanza di questi princìpi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità. Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 luglio 1995, n. 345, ha chiarito che l'attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini, come invece questo disegno di legge Riteniamo che, se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, ossia la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l'imposizione di un'esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto. L'iscrizione all'albo degli avvocati - come abbiamo detto anche in fase di discussione generale - non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l'esclusiva. La necessaria presenza di un avvocato nella veste del difensore, anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative, a nostro modo di vedere, rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò dì vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile. In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente, secondo noi, le conseguenze negative dell'eventuale approvazione del disegno di legge legge qualora non dovesse venire emendato nella direzione in cui molti Gruppi dell'opposizione hanno presentato degli emendamenti. L'estensione degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determina altresì una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale. Ringrazio per l'attenzione e rinnovo ancora una volta l'invito alla partecipazione attiva alla difesa degli emendamenti perché mi par di capire che in alcune circostanze, poc'anzi, la partecipazione stessa ha contribuito a far mutare in corso d'opera alcuni dei pareri del relatore e del Governo.

alla possibilità che uffici legali di associazioni di categoria e sindacati svolgano attività di consulenza. Tutto questo è contemplato nell'emendamento 2.245, ma non condivido la possibilità, che lui adombrava, che ex dipendenti di queste associazioni ed enti possano, una volta concluso il rapporto di lavoro, continuare a svolgere attività di consulenza legale, perché sarebbe un modo surrettizio anche per dribblare quelle procedure di approdo all'attività di avvocato attraverso una serie di scuole di specializzazione, concorso, abilitazione e così Quindi, chiaramente, si potrebbe costituire una seconda via che darebbe anche meno certezze di qualificazione.

Presidente, ho presentato il solo emendamento 2.226, che riguarda i commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Senatore Valentino, il senatore Pastore sta richiamando la sua attenzione.

da qualche collega dell'opposizione degli «avvocati fai da te», improvvisati, che assumono una difesa in giudizio con scarsa o nulla esperienza e che quindi incappano sicuramente nei trabocchetti non solo delle norme sostanziali ma in quelle ma in quelle di procedura, che sono altrettanto delicate quanto le norme sostanziali. Invece ho una visione assolutamente conforme a quella del disegno di legge tant'è che il comma 5, che io riscrivo, tende ad evitare un equivoco, cioè che la deroga all'esclusiva degli avvocati nell'esercizio della difesa possa riguardare la stessa funzione dell'avvocato. Se il relatore legge il comma 5, così com'è stato scritto nel testo del disegno di legge, «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge

La mia riformulazione tende invece a confermare che comunque all'avvocato compete il diritto di difesa in via esclusiva salvo che l'esclusiva sia modificata dalla norma di legge. la riscrittura del comma 6, che riguarda la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale. Così com'è formulata, la norma può indurre a ritenere che solo in caso di espresse previsioni di legge questa consulenza non possa essere formulata da altri soggetti, sia professionisti, sia titolari di funzioni alle quali si riconosce una certa autorevolezza in materia giuridica. Faccio l'esempio, anche nel corso del dibattito, dei professori universitari in materia giuridica, i quali magari non sono iscritti all'albo degli avvocati e che sono chiamati spesso a spesso a formulare e sottoscrivere pareri *pro veritate* che sono vere e proprie forme di consulenza legale. Mi riferisco anche ad altre figure professionali che

Credo che si tratti di una questione estremamente delicata. Non ritengo che il diritto comunitario abbia liberalizzato tutto, né che le professioni siano equiparabili all'attività di impresa, né che il sistema ordinistico sia ripudiato o sia lontano dai modelli europei: anzi, è accettato ed è ben presente non solo in Italia. Però mi preoccupano certe formule legislative che possono, nell'ambito di categorie che svolgono attività di questo tipo, apparire troppo radicali, e quindi mi permetto di formulare questo emendamento, naturalmente augurandomi che il relatore e il Governo possano trovare una soluzione a questo che è uno dei problemi più acuti e più specifici dell'elencazione delle attribuzioni all'avvocatura. È chiaro che l'avvocato ha competenza ampia ed illimitata proprio per la formazione che ha,

che imprese, associazioni e altri enti o istituzioni, in virtù dell'articolato attuale, non possano più continuare a prestare assistenza e consulenza legale a beneficio dei propri associati, ed è per questo che

Una consulenza altamente professionale, pur rimanendo consulenza e pur rimanendo occasionale, secondo tutte le statistiche è di qualità nella misura in cui essa viene richiesta da molti. Anche quella prestazione occasionale deve essere allora concessa perché tale non rimarrà, ma diverrà di largo utilizzo.

fine, la seguente formulazione: «È fatta salva la possibilità di svolgere consulenza legale per i professori universitari di materie giuridiche laureati in giurisprudenza».

con la seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti». Tutta la parte iniziale, ossia «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione»,

210 iniziano a sollecitare l'attenzione su questa riserva dell'attività dell'avvocato.

di cui ai commi 5 e 6. 2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società

mi chiedo cosa dovranno fare gli avvocati di domani per essere una sorta di paladini di un mondo più giusto in cui tutto va bene.

poco fa e che interessano leggi approvate da poco. In particolar modo, ci si riferisce a tutte quelle attività di conciliazione, di mediazione, che servono molto servono molto a snellire l'apparato della giustizia, ma inserendo le parole «in ogni sede» in realtà si mette un'ipoteca su quelli che saranno invece compiti solo ed esclusivamente dell'avvocato.

un avvocato. Di citazioni ne abbiamo già fatte altre in merito a direttive europee. In questo caso, cito maggio 2006 della Cassazione che riprendo dal *dossier* del Servizio studi del Senato, in cui testualmente si dice: «La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, comunque di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli

«l'iscrizione ad un albo circondariale», bensì «il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 46». Questo, secondo noi, va ancora una volta a tutelare

ai magistrati o ai docenti universitari di materie giuridiche di accedere all'albo professionale se non attraverso un esame mi sembra in qualche modo surreale. il quale siamo in attesa del parere della Commissione

voto favorevole. Desidero sottoporre all'Aula il seguente problema. Si tratta, in sostanza, della possibilità per i professori universitari in materie giuridiche di essere iscritti di diritto nell'albo degli avvocati. Credo che ben cinque argomentazioni depongano in favore di questa normativa, che è quella vigente e che il disegno di legge chiede invece di abrogare. universitario in materie giuridiche contribuisce ad esaminare il futuro avvocato e fa parte della commissione di abilitazione per l'avvocatura.

Ho capito che c'è un ostruzionismo di maggioranza e di minoranza.

in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Questo è un tema che negli ultimi tempi è stato particolarmente sentito e analizzato da più parti dell'avvocatura e dalle varie anime associative, sia in sede penale che in sede civile. Per questo motivo molti ordini forensi, per esempio i comitati pari opportunità, hanno avvertito la necessità e l'esigenza di giungere alla sottoscrizione di protocolli d'intesa che fossero utili strumenti per l'attuazione del principio di parità di genere e per la rimozione di disparità di trattamento in ambito legale. Questi documenti, recepite le esigenze che si sono manifestate nelle varie componenti dell'avvocatura, si sono dimostrati idonei per promuovere tra tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati) ogni iniziativa necessaria per la sensibilizzazione sui temi dell'astensione dell'avvocato donna per il periodo corrispondente al congedo di maternità. Bisogna ricordare che la donna avvocato, come libera professionista, non vede assolutamente garantito e tutelato il diritto alla maternità, come avviene invece per le

in questo senso, perché evidentemente si tratta di tutelare il diritto dell'avvocato donna all'esercizio della professione, nel rispetto ed in attuazione degli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione.

CEE, come modificato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; a numerose direttive che riguardano l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione; alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

tra tutte quelle di genere, obiettivo primario che l'Unione europea si è data in questi ultimi anni. Quindi, un'azione positiva atta e finalizzata alla realizzazione della parità tra i generi. Nella professione forense si è sentita e si sente fortemente la necessità di recepire queste disposizioni per attuare misure di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, dando in questo modo il via alla costituzione dei comitati pari opportunità presso gli ordini forensi, organismi paritetici con funzioni consultive e di promozione delle politiche di azioni positive. Concludo dicendo che, sulla base delle problematiche emerse da un recente

che ha tenuto conto del ruolo di cura e del necessario bilanciamento di questo ruolo con le esigenze di una professione sempre più competitiva, uno dei principali compiti che la commissione pari opportunità del Consiglio forense ha ritenuto di avere è stato proprio quello di suggerire la produzione di questo emendamento, con un testo in linea con la normativa nazionale e sovranazionale indicata. Il tema quindi è di particolare importanza e non può essere sottovalutato. Lo stesso relatore ne ha convenuto per quanto riguarda il merito dell'emendamento

formulo un ordine del giorno impegnativo per il Governo affinché alla prima occasione utile si possa rendere giustizia ad un mondo importante, superiore a quello

espressioni cui corrisponda sempre un senso univoco. Se il relatore vuole specificare da che cosa si intende esentare l'avvocato con questo comma, potremmo valutare il senso della norma; se, invece, non c'è risposta su questo punto,

soggetti al contratto; in proposito posso soltanto ricordare che il contratto è disciplinato secondo la legge, per cui è sempre la legge che disciplina il contratto. Parimenti, il codice deontologico è fissato per legge o per norma secondaria, per cui l'espressione contenuta all'articolo 2, comma 4, ha una sua ragion d'essere, perché rispetto della legge significa rispetto anche dei contratti da essa disciplinati, nonché rispetto della deontologia, che è disciplinata dalla legge o da norma secondaria.

può assumere ogni determinazione ed è soggetto esclusivamente alla legge,

**Il Senato non approva**.

*(PD)*. Mi pare che sia contraria ai criteri di economicità e di comprensibilità delle votazioni, ma non

Presidente, abbiamo nel nostro ordinamento - credo - un unico precedente di una disposizione che indica la soggezione di una categoria soltanto alla legge. Questo precedente è l'articolo 101 della Costituzione, che per la sua collocazione sistematica ha un significato: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». un'affermazione di grande significato in un sistema - quello costituzionale italiano - che adotta la separazione dei poteri e il sistema complesso di controlli incrociati e di reciproche autonomie come una delle caratteristiche fondamentali dell'ordinamento repubblicano democratico. Il fatto di ribadire in una legge ordinaria che gli avvocati sono soggetti soltanto alla legge non ha nessun significato, se non quello di una replica in tono minore. Mi lasci dire che è anche alquanto inadeguato inadeguato al valore, alla funzione e alla dignità sociale della professione di avvocato introdurre questo principio a tutti i costi, magari sperando che un giorno o l'altro se ne possa avere, grazie ad un legislatore distratto, anche una versione di natura costituzionale. una versione di natura costituzionale. Messa così, questa previsione non ha assolutamente alcun senso. Ho ascoltato con molta attenzione l'argomentare del senatore Longo e mi è sembrato un ragionamento tautologico che non portava da nessuna parte. Ho ascoltato con altrettanta attenzione l'intervento del professor Ichino e mi sono pienamente convinta, a questo punto, della ragionevolezza dell'emendamento che avevamo presentato e che l'Aula ha invece respinto. La ragione è semplice: qual è questo potere di fronte al quale, peraltro con legge ordinaria, bisognerebbe ribadire la soggezione dell'avvocato soltanto alla legge? È davvero un *nonsense*

Attribuisco un'altra interpretazione, e per questo chiedo al collega se può preliminarmente dare un chiarimento: o questo questo comma - e quindi la circostanza che si dica che nell'esercizio della propria attività l'avvocato è soggetto solo alla legge - è una cosa ovvia, tautologica (chiamiamola come vogliamo: mi sembra anche questa estremamente surreale)

la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, l'organizzazione del funzionamento degli organi professionali e quant'altro, non è soggetta all'esercizio del potere normativo

insieme a un problema legato all'ammissibilità dell'emendamento, cioè la mancanza di emendamenti conseguentemente soppressivi, perché ogni parte del testo in cui si attribuisce alla fonte normativa secondaria (regolamento) di disciplinare alcune attività

Sono certo che l'emendamento soppressivo del comma 4 non è passato in Aula: quindi adesso il testo è quello originale, che recita: «Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'Ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge». Se viene respinto l'emendamento Caruso, tautologicamente, rimane in vita l'attuale comma 4 dell'articolo 2. Non vi è dubbio: sarà banale, ma è così.

questi emendamenti. Ho sommessamente detto che anche a me il comma 4 dell'articolo 2 sembrava una non utile parafrasi della norma costituzionale che riguarda i magistrati. Ma il senatore D'Alia sa, come so io, che, come si usa dire, «piuttosto che niente meglio piuttosto». Di qui l'emendamento a esito non fortunato che precede questo, che voleva distinguere tra coloro che svolgono funzioni nel contesto della professione - quindi, gli ordini ed il Consiglio nazionale - e l'avvocato nella sua attività, in esame è la subordinata della subordinata sul piano logico e sul piano sostanziale, in quanto si limita all'avvocato e alla sua attività. Per il resto, rimando a quello che dice il senatore Longo: se è preferibile il testo nella sua nella sua ipertrofia originaria, basta respingere l'emendamento ed il risultato è conseguito.

introduce una specificazione superflua. Stiamo approvando una legge che organizza e disciplina l'esercizio dell'attività forense e, quindi, il riferimento alla soggezione soltanto alla legge deve intendersi alla legge dell'ordinamento professionale, o è un riferimento generico alla legge? Il riferimento generico alla legge non è necessario, mentre il riferimento alla legge professionale, se è questa la legge professionale che disciplina l'attività, diventa inutile. Il problema è che nel testo attuale è è inserito, con una collocazione impropria (è un errore tecnico), anche l'ordine professionale, che invece è disciplinato all'articolo 23.

all'avvocato (cioè ai soggetti) e non all'Ordine forense, che ha un'altra collocazione sistematica nel disegno di legge. Ha quindi più senso

mi scuso perché in realtà non avevo ascoltato la sua illustrazione. Tuttavia, devo dire che è stato ancora più illuminante e decisivo per il nostro voto contrario su questo emendamento l'intervento del senatore Longo, molto preciso e puntuale nella sua spiegazione, che porta al seguente risultato: non alla circostanza, senatore Li Gotti, che l'avvocato resti sottoposto alla legge nella sua attività quanto alla circostanza che si riconosce, con l'esclusione degli ordini una autonomia normativa e organizzativa agli ordini professionali forensi a prescindere dalla legge. così, senatore Longo, perché nel momento in cui il testo finale prevede che l'Ordine forense non è più sottoposto alla legge salvo tutto ciò che viene fatto e che è ricompreso nell'ambito delle fonti previste, per il resto valgono i principi costituzionali e la disciplina in materia di autonomia

che non siano in conflitto con la legge e quindi con le competenze che sono riservate dalla legge anche alla potestà normativa, e si prevede che vi sia una fonte ulteriore di produzione normativa per quanto riguarda l'attività forense. Questo è il risultato finale che, secondo me, all'esito dell'eventuale accoglimento dell'emendamento del senatore Caruso, ci troveremo di fronte. Per queste ragioni, il voto del mio Gruppo sarà contrario.

che testualmente prevede l'esclusività dell'avvocato per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali (e ovviamente non sarebbe questo il problema), ma anche nelle procedure arbitrali rituali (sul punto poi interverremo anche con un altro emendamento). Il problema più in generale riguarda questo continuo riconoscere soltanto all'avvocato la possibilità di assistere la persona che ne ha bisogno e difenderla nei vari giudizi. In realtà, ricordo che l'ordinamento italiano conosce e regola fattispecie rilevanti di deroga tale riserva di attività; persino nell'ambito della difesa e della rappresentanza in giudizio, in tutte le ipotesi che poi elencherò, le parti, siano esse privati o pubbliche amministrazioni, possono stare in giudizio senza difesa tecnica. A mero titolo esemplificativo, basti ricordare le sanzioni amministrative, il contenzioso tributario, le cause civili ordinarie dinanzi al giudice di pace in materia di contenzioso del lavoro delle amministrazioni pubbliche. Insomma, c'è

che è il mercato della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale: riducendo il numero dei commensali la fetta aumenta per chi è rimasto a tavola, ovvero gli avvocati iscritti all'Ordine. Ciò può avere un senso dal punto di vista economico di chi rimane seduto a tavola,

e, quindi, a possibili procedure d'infrazione e a tutto un *iter* complicatissimo che sicuramente non garantirà la certezza del diritto. Il legislatore ha facoltà di esigere qualsiasi titolo o condizione legale per l'esercizio di qualsiasi attività, attività, ma gli è vietato introdurre dei limiti alla libertà di concorrenza e, poiché in altri Paesi europei non esiste (lo abbiamo citato prima) la riserva di assistenza stragiudiziale all'ordine forense, è ragionevole sostenere che questa riserva, anche ad ammettere l'idea di inserirla in una legge, non può essere assoluta e inderogabile. La riserva di attività non può avere la funzione di proteggere una categoria professionale dalla concorrenza concorrenza (in questo caso la norma si porrebbe in contrasto con il Trattato e con l'Unione europea), ma solo quella di aumentare il tasso di professionalità esigibile da chi deve svolgere attività a favore del pubblico, pubblico, di consumatori e utenti, a maggiore garanzia di questi ultimi. L'esistenza degli ordini viene ammessa dalle leggi laddove questi ordini tutelino

sindacati di vario tipo si sono vantati di avere tesserati falsi e, quindi, anche i sindacati e i patronati che daranno consulenza legale

della sua forza nella riformulazione, mi comporterò di conseguenza anche sull'emendamento interamente soppressivo, che non voterei se invece l'emendamento

mi pare di aver capito che si tratta di una riformulazione che ingloberebbe anche un precedente emendamento riformulato, per il quale siamo in attesa del parere della Commissione bilancio. Pertanto, per capire esattamente qual è la portata di questo testo, prima di votarlo, chiederei la cortesia, cortesia, non solo a nome mio, ma anche degli altri colleghi, di poter leggere il testo e valutare se non debba anch'esso essere sottoposto al parere preventivo della Commissione bilancio. la Presidenza fa una proposta. Dopo aver innanzitutto confermato al senatore D'Alia che la Presidenza ritiene che la nuova formulazione vada comunque sottoposta alla Commissione

come segue: «L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato». Secondo me, esiste al riguardo un problema di fondo e più interessante relativo all'Ordine degli avvocati.

la condizione prioritaria era quella di essere iscritti ad un albo circondariale. Con il comma 7 si va oltre e si specifica che perfino l'uso del titolo dipende non tanto dalla laurea, dal

Fa specie che lo si possa conservare anche quando non si è più iscritti all'albo, che è la condizione per esercitare la professione.

sostenendo che gli Ordini, in realtà, non devono essere degli enti pubblici obbligatori, ma appunto quello che in realtà sono, vale a dire dei soggetti privati che tutelano gli iscritti e

perché credo sia corretto che chi non eserciti la professione non si possa fregiare del titolo,

a fine carriera, non capisco la ragione per la quale stiamo facendo tutta questa discussione su come chiudere - e non su come selezionare - l'accesso alla professione per poi - l'accesso alla professione per poi dire che chi, ad esempio, è cancellato dall'albo perché non ha la continuità dell'esercizio professionale comunque

la soppressione debba essere letta nel contesto e unitamente all'articolo 20 del disegno di legge.

ossia della persistenza del titolo, vale a dire della possibilità di utilizzo del titolo di avvocato anche quando si sia stati iscritti. Essere stati iscritti ad un Albo un qualcosa di concreto, di specifico e di articolato, che è disciplinato dall'articolo 20. Se si parte da tale articolo si capisce anche questa norma. Sicché ritengo che la previsione del comma 7 sia corretta e voterò contro l'emendamento.

consulenze avrebbero potuto essere date solo agli iscritti o agli associati di una determinata organizzazione che si ritiene siano parte di quell'associazione nel momento in cui viene fornita la consulenza. Qui addirittura si vuole iscrivere nella casta - perché si sta veramente creando una casta - degli avvocati coloro i quali sono stati iscritti, ma oggi potrebbero non esserlo più. In conclusione, non soltanto dichiaro il voto favorevole, ma chiedo anche la votazione con il sistema elettronico.

sono lieta di accogliere un ordine del giorno che, anche attraverso lo strumento degli studi di settore, propone di offrire un aiuto concreto alle donne nell'espletamento della loro attività professionale. Tutti sanno che le donne spesso si trovano nella difficoltà di dover svolgere un doppio ruolo, ruolo, quello che riguarda l'attività domestico-familiare e quello che riguarda l'attività professionale. Quindi, sarebbe assolutamente penalizzante ed ingiusto che a questa difficoltà si aggiungesse poi anche una valutazione sotto il profilo

precisamente quello di ottenere, per le avvocate che svolgono individualmente la libera professione e per tutte le professioniste nelle stesse condizioni, che l'anno in cui c'è stata gravidanza o una situazione ad essa assimilata sia, al fine degli studi di settore, adeguatamente considerato perché è ovvio che in quell'anno il reddito è assolutamente diverso. Riteniamo quindi che questo impegno del Governo sia sufficiente. Specifico al riguardo

da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008***

Signora Presidente, vorrei cogliere l'occasione dell'esame di questo Trattato per osservare come la Commissione esteri sia riuscita negli ultimi tempi ad esaminare e definire, anche congiuntamente ad altre Commissioni, un gran numero di accordi internazionali, il che ha permesso di recuperare i ritardi nell'adempimento di fondamentali obblighi internazionali assunti negli anni dal nostro Paese. Ciò è stato possibile grazie allo spirito di leale collaborazione tra le forze politiche, tra maggioranza ed opposizione, di cui voglio qui dare atto ai colleghi. In più di un'occasione, peraltro, la Commissione ha esaminato i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica promossi da singoli parlamentari, anche dell'opposizione,

rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione dei Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità sono la stabilizzazione della situazione politica,

sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale della regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; intensificare la cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione, stante anche la situazione più avanzata della Croazia. Con l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea. altri Accordi, che l'erogazione dell'aiuto comunitario sia subordinato al conformarsi ai criteri politici di Copenaghen ed all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche.

Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo Accordo di stabilizzazione, che è l'ultimo che le Comunità europee stipulano con i Paesi dei cosiddetti Balcani occidentali. La Bosnia-Erzegovina è un Paese che è stato tenuto sotto tutela internazionale fin dalla Conferenza di Dayton del 1995, sulla quale più volte ci siamo soffermati circa gli esiti non necessariamente positivi. Tra quelli sicuramente negativi c'era il fatto di aver convocato Slobodan Milosevic al tavolo di coloro i quali avrebbero dovuto assicurare la pace in quella parte del mondo, pace che lo stesso Slobodan Milosevic Slobodan Milosevic ha continuato a calpestare fino a tutto il 1999. La Commissione europea nel 1999 aveva, in effetti, avviato i negoziati di questo patto di stabilità e credo che nessuno più di lei, signora Presidente, fosse coinvolto in quel tipo di iniziativa, vista e considerata la sua sensibilità nei confronti della pace da perseguirsi attraverso l'affermazione della giustizia internazionale in tutti i Balcani. La ratifica di questo

all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) perché si avvii un processo di de-etnicizzazione del Paese: è una questione fondamentale, visto e considerato che la ratifica dell'Accordo che ci apprestiamo a votare tra poco

le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007*** «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: la Commissione, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per le altre ratifiche, recanti identica copertura, già presentate alle Camere e non ancora discusse.».

Il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, delinea un processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona.

Il primo è che questa Dichiarazione di intenti è stata firmata dal ministro Martino nel 2004 e nel 2007 dal ministro Parisi. Quindi, è un trattato che parte da lontano; anticipa in effetti il Trattato di Lisbona ed inizia a mettere insieme un rafforzamento della politica europea di sicurezza e di difesa. La seconda valutazione che vorrei sottoporre ai colleghi è riferita al fatto che l'Arma dei carabinieri è la forza che rappresenta l'Italia in questo dispositivo di sicurezza

proprio perché viene da lontano e perché ha avuto tempi lunghi, abbiamo ritenuto, anche con la disponibilità in particolar modo del sottosegretario Crosetto,

Il secondo punto oggetto dell'ordine del giorno è la questione della garanzia per quanto riguarda la partecipazione ed il controllo democratico da parte dei Parlamenti nazionali, UEO ha esaurito la sua missione ed i suoi compiti; pertanto tale materia rientra nelle competenze dell'Unione europea e quindi si pone il problema del controllo dei Parlamenti nazionali e anche del Parlamento europeo. Il terzo impegno che chiediamo al Governo è quello di provvedere ad un riordino delle voci di bilancio proprio per garantire questa partecipazione forte ed efficace dell'Italia alla costruzione della politica europea di sicurezza e difesa comune.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Grazie, Presidente. la positività del contenuto di questo provvedimento era emersa anche in sede di Commissione, dove ha trovato parere fortemente e convintamente favorevole da parte di tutti i Gruppi. È un onore per me far presente che è stato scelto come quartier generale la caserma Chinotto, attuale scuola allievi dei brigadieri dell'Arma, di Vicenza, la mia città, e quindi ricordare anche che il comando spetterà ai Carabinieri. L'istituzione di questa nuova forza testimonia che le Forze armate italiane possono essere evidentemente protagoniste in ambito europeo

è quello in parte accennato nell'ordine del giorno della senatrice Marinaro e cioè che qui si sta facendo l'economia di quella che è diventata l'Unione europea. Credo in modo particolare che tutte le volte che si va a creare una cooperazione intergovernativa si diminuisca lo spirito che invece dovrebbe essere al centro dell'Unione stessa, cioè quello di far diventare quanto più europeo possibile tutto ciò che coinvolge Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di specie, essendo da sempre il Partito radicale a favore della smilitarizzazione della polizia credo ci sia un ulteriore argomento. L'altro motivo per cui non parteciperò al voto è il terzo il terzo impegno che ha preso il Governo oggi, cioè il finanziamento di tale provvedimento. Si vanno a distrarre fondi da ciò che era stato accantonato per la lotta alla desertificazione.

internazionali avevano a tutt'altri fini indirizzato, comunque fondamentali per il mantenimento anche della pace e della sicurezza in buona parte del mondo, credo non si possa partecipare ad un voto favorevole.

grande rilievo a una conferenza stampa tenuta ieri dal sottosegretario Bertolaso, nonché capo della Protezione civile, sull'emergenza vulcani in Italia. La conferenza stampa probabilmente era collegata all'allarme, e anche alla tragedia, derivante dalle eruzioni in Islanda, ma il Sottosegretario ha fatto il punto sulla questione dei vulcani in Italia e lo ha fatto, lo ha fatto, lo dico eufemisticamente, con improvvide frasi, anche un po' colorite, che però, riguardando invece situazioni serie come quella del vulcano Vesuvio Vesuvio e del monte Epomeo ad Ischia, hanno suscitato un indicibile allarme. Il Sottosegretario ha usato una frase molto colorita e cioè che l'isola di Ischia ha il «colpo in canna» da fucile armato. Sono frasi che, tra l'altro, nella giornata di oggi sono state smentite da molti esperti in materia di vulcanologia, ma che tuttavia, signora Presidente, hanno suscitato un giustificatissimo allarme, tanto per cominciare in chi ha il dovere di sovrintendere alle questioni locali, cioè i sei sindaci di Ischia, che giustamente hanno chiesto un immediato incontro - che noi sosteniamo - con il Sottosegretario affinché spieghi, magari in una riunione in cui ci siano anche degli esperti e in cui si possa fare sulla materia un approfondimento scientifico,

Nel testo del rapporto, che oggi è stato reso noto, vengono analizzate sette operazioni condotte fra il 6 maggio e il 31 luglio 2009, con destinazione Libia e Algeria. Ecco la descrizione che viene fatta di alcune di tali operazioni: i migranti sono stati lasciati sul ponte di una nave con poca acqua, senza cibo, né coperte anche per 12 ore, dopo un viaggio durato giorni che li ha lasciati disidradati, in stato confusionale e, alcune volte, in stato comatoso. Tra loro potenziali richiedenti asilo, o persone che hanno ricevuto documenti temporanei dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma anche minori e donne in avanzato stato di gravidanza. In alcuni casi, hanno subìto maltrattamenti tali da dover essere ricoverati, oppure si sono visti togliere tutti i loro beni senza che gli fossero mai restituiti.

La richiesta, avanzata oggi all'Italia dal Comitato per la prevenzione della tortura, è che tutte le persone sotto la sua giurisdizione ricevano le necessarie cure mediche e l'assistenza umanitaria che il loro stato richiede, in modo che abbiano accesso alle procedure in grado di garantire il rispetto del diritto di non respingimento. suddetta richiesta se ne aggiunge anche un'altra, recente, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, affinché si risponda sui respingimenti collettivi dei migranti verso la Libia. Ricordo altresì che, in risposta a un'interrogazione parlamentare presentata insieme alla senatrice Poretti relativamente agli accordi ulteriori stipulati con il Governo del colonnello Gheddafi, ci è stato risposto che nessuno dei quattro accordi ha a che fare con materie attinenti all'immigrazione. Desideriamo pertanto sapere,

Domani, qui a Roma, ci sarà finalmente l'incontro tra il ministro Scajola, il vice ministro Romani e le rappresentanze sindacali dell'Italtel, che in modo sorprendente ha disdetto unilateralmente l'accordo relativo ai contratti di solidarietà. di un'azienda che rappresenta l'eccellenza nelle comunicazioni, con una struttura di circa 1.970 dipendenti in Italia; a Carini, una cittadina dell'*hinterland* palermitano dove insiste un'area industriale, i dipendenti sono 225, di cui 170 ricercatori. Il Governo Prodi aveva stanziato dei fondi per la banda larga, che sono stati gestiti dal Governo Berlusconi, e metà di essi sono stati destinati all'Abruzzo. Per il resto non si sa nulla. Mi auguro che l'incontro di domani sia foriero di risultanze significative. Qualora non si dovessero dare risposte adeguate, il Governo sarà ancora una volta agli annunci prima e alle bugie dopo di fronte a un aumento della disoccupazione in Sicilia che, nonostante la